Sono di oggi le parole allarmate di Jean Claude Trichet: «La crisi del debito ha ormai raggiunto dimensione sistemica e nelle ultime tre settimane è peggiorata». Vi è da parte vostra una sorta di diserzione, che è etica prima che politica, dai doveri del governo di una Nazione in tempo di crisi. Ci sono i dati drammatici del PIL. Dice il Governo: «Rispetto al Documento presentato ad aprile si ipotizza una minore crescita cumulata sull'orizzonte previsivo pari a circa due punti percentuali. Fuori dall'Italia, nell'economia internazionale, si manifestano purtroppo analoghi andamenti negativi». Andamenti negativi certamente, ma analoghi non possiamo dirlo, visto che la crescita in Eurolandia è comunque stimata dal Fondo monetario internazionale all'1,4 per cento, il doppio dell'Italia. Al 2014, l'Italia, con ritmi di crescita di qualche decimo di punto all'anno, non avrebbe neppure recuperato la ricchezza perduta nel biennio 2007-2008. Un Paese fermo ed un Governo fermo: è questo che non possiamo permetterci e che rende insostenibile nelle valutazioni degli analisti il nostro debito. l'incapacità politica di creare una successione ad un Presidente del Consiglio screditato nell'opinione pubblica italiana ed internazionale; l'incapacità tecnica, e insieme politica, di predisporre ed approvare provvedimenti capaci di orientare il Paese su un sentiero di maggiore crescita. È dall'inizio dell'anno che il Governo promette provvedimenti per la crescita. Ricordiamo la famosa frustata per l'economia che avrebbe prodotto una crescita mai vista: era la conferenza stampa del gennaio scorso del Presidente del Consiglio. Da qualche settimana si promette un decreto per lo sviluppo, rinviato di giorno in giorno. Capiamo che mancano le idee, manca una visione del Paese, manca il coraggio di riforme vere e, da quanto apprendiamo sulla stampa, si sta ripiegando sulla viltà politica ed etica dei condoni. Si registra una elevata pressione inflativa, destinata ad essere incrementata dall'aumento di un punto dell'IVA che si sta trasferendo sui prezzi dei beni finali in misura ben superiore.

(non a caso, mercati a scarsa concorrenza). Al 2013, più di otto decimi della modesta crescita sarebbero dovuti alla domanda interna, essendo il contributo dell'*export* limitato a un modesto 0,1 ma, con un'inflazione in crescita e senza sviluppo e mancati interventi di sostegno della domanda, è possibile che neppure questo modesto *target* possa essere raggiunto. La pressione fiscale raggiungerà il record del 43,9 per cento del PIL, il valore più elevato da quando esiste la Repubblica italiana. Cari colleghi della Lega, questo è il vostro contributo al governo della Nazione: la pressione fiscale più elevata dal dopoguerra, ma anche la più iniqua, perché ciò che è stato fatto e ciò che ci si è impegnati a fare accresce l'iniquità del sistema fiscale. I propositi di lotta all'evasione sono già indeboliti solo dal fatto di parlare di nuovo di condoni. Si fanno annunci e non si fanno le cose semplici. Il documento «Progetto delle imprese per l'Italia», firmato dalle principali associazioni del mondo imprenditoriale, riprende le proposte formulate dal Partito Democratico: eliminazione del contante per le transazioni sopra i 500 euro. Uno studio dell'ABI stima che, se vi fosse una diffusione in Italia dei pagamenti con moneta elettronica pari alla media europea (oggi siamo poco sopra la metà), si realizzerebbe un recupero di evasione fino a 30 miliardi di euro. Ecco le riforme senza oneri. È noto che il complesso delle due manovre, quella di luglio e quella di settembre, si finanzia per il 73 per cento con maggiori entrate, accrescendo l'iniquità del sistema percentuale è destinata di fatto ad aumentare se si tiene conto del fatto che il taglio della finanza locale, che tocca spese obbligatorie, dovrà essere affrontato con un aumento della pressione fiscale a livello locale. L'avvio dell'esame della delega fiscale alla Camera dei deputati ha già fatto emergere una stroncatura sul piano tecnico, per errori materiali, per contraddizioni con i decreti sul federalismo, per l'indeterminatezza della delega: prevedere tre aliquote e non fissare gli scaglioni significa non dire nulla, o meglio una sola cosa, che comunque gli unici sicuramente avvantaggiati saranno i redditi superiori ai 75.000 euro annui. della delega comporterebbe un innalzamento intollerabile dell'iniquità fiscale. Al 2014 si dovrebbero ricavare 20 miliardi dalla revisione della spesa sociale ed assistenziale e dalla revisione dei regimi fiscali agevolativi. Ora, la spesa di competenza statale per il sociale ammonta a 30 miliardi di euro, e si chiama assegni familiari, assegni per l'invalidità e assegni sociali. Si potranno combattere gli abusi, ma certamente non si ricaveranno cifre significative. Vi concentrerete necessariamente sui regimi fiscali agevolativi, e sono interventi essenziali per la tenuta dei bilanci familiari dei redditi più deboli. cento degli importi delle agevolazioni riguarda detrazioni per il lavoro dipendente e le pensioni, per i carichi familiari, per le spese sanitarie e di studio, per i mutui casa; interventi agevolativi sull'IVA e sulle accise: beni di largo consumo e riscaldamento. L'attuazione della delega così come impostata comporterebbe una drammatica correzione regressiva del sistema fiscale. Il peso si distribuirebbe con un accanimento inconcepibile sui redditi bassi e nulla verrebbe chiesto ai redditi e ai patrimoni più elevati. Infine, gli investimenti: rispetto al 2009, la spesa in conto capitale risulta dimezzata; già ai livelli minimi nel 2009, scende al punto di non consentire neppure modestissimi programmi di manutenzione. Prendiamo come eravamo nel 1997: anche allora una manovra difficile, fatta da un Governo responsabile per agganciare l'euro, eppure allora, per ogni 100 euro per le spese correnti, se ne investivano 15 in conto capitale. Oggi, per ogni 100 euro di spesa corrente, ce ne sono solo 5 di investimenti, in un Paese con un drammatico *deficit* infrastrutturale e di manutenzione del territorio. La velocità media di connessione Internet è in Italia di 3 megabit al secondo, la metà della Romania. Siamo indietro sulle infrastrutture tradizionali della logistica (porti e ferrovie in particolare) e abbiamo già accumulato un ritardo vergognoso su quelle innovative. Bisogna non solo ridurre la spesa, ma cambiarne profondamente il *mix*. E' molto difficile, certo: basti pensare che nell'ultimo decennio, a fronte ad un aumento del totale della spesa delle amministrazioni centrali del 27 per cento, la spesa pensionistica è aumentata del 47 per cento e quella sanitaria del 51 per cento. Bisogna agire, ma si può agire in due settori così delicati dal punto di vista dei diritti fondamentali solo avendo la bussola dell'equità e della giustizia sociale: riferimento totalmente mancato nella politica economica del Governo. Nel concludere, signora Presidente, sottolineo siamo puniti dai mercati, che molto lavorano sulle aspettative. Perché la Spagna in giugno aveva uno *spread* sui titoli tedeschi peggiore del nostro di 70 punti, e oggi questo *spread* è migliore di 40 Nulla è cambiato sui fondamentali dell'economia e della finanza, solo che lì c'è un Governo che governa anche alla soglia delle elezioni e che costruisce intese con l'opposizione, invece di insultarla. Qui c'è un Governo che "sgoverna", che ignora un'agenda di crescita, che è senza il sostegno delle parti sociali, che divide il Paese e la politica, aggrappato ad un potere che non sa più gestire. Paghiamo la «papi *tax*» di cui ha parlato l'economista Tito Boeri. Il Paese non può più sopportarla.

come già il Documento di economia e finanza, esaminato solo pochi mesi fa, nel mese di aprile, la Nota di aggiornamento oggi all'esame costituisce la prima applicazione del nuovo ciclo di programmazione economica e finanziaria delineato della legge n. 39 del 2011, che ha modificato la disposizioni della legge di contabilità e finanza pubblica, al fine di dare attuazione nel nostro ordinamento ai cosiddetto semestre europeo. Quanto al contenuto del documento all'esame dell'Assemblea, i dati mettono in rilievo la perdurante difficoltà della situazione economica nel nostro Paese. Il dato di sintesi, forse di maggiore interesse, sta nella minor crescita che l'economia italiana sperimenterà nel periodo 2011-2014, rispetto alle previsioni originarie del DEF: una crescita complessiva e cumulata, prevista in circa 2 punti percentuali, spalmata negli anni dal 2011 al 2012 fino al 2013, quando risale di poco, all'1 Confrontando un simile percorso in risalita del PIL con il dato della caduta della crescita, quello del 2009 - ricordiamolo tutti - a meno 5 per cento, risalta chiaramente la complessità della situazione in cui il nostro Governo deve operare. È giusto, però, anche ricordare come l'andamento di alcuni dati (per esempio, quelli sull'occupazione e sull'*export*) siano in controtendenza e facciano già registrare timidi segnali positivi di ripresa.

signora Presidente, cerco di portare via meno tempo possibile ai lavori dell'Aula. Ritengo utile il confronto con i dati dell'economia americana, risultata di un terzo inferiore

dei Paesi emergenti, che, dalla previsione del 6,3 per cento, scendono al 5,9 per cento. Il rallentamento dell'economia globale e il riemergere delle tensioni sui mercati finanziari, e, in particolare, sul debito sovrano dei Paesi dell'area dell'euro, hanno determinato, nel complesso, un deterioramento delle prospettive di crescita dell'economia globale. Da un lato, quindi, la Nota di aggiornamento presenta questa revisione del quadro macroeconomico - e non avrebbe potuto che essere così e, dall'altro, il documento oggi all'esame evidenzia come, per fronteggiare la difficile congiuntura economica e finanziaria, europea e mondiale, sia stato necessario intraprendere un percorso accelerato di approvazione delle manovre correttive di finanza pubblica, che non ha non ha potuto quindi seguire integralmente il calendario scandito dalla legge e dal semestre europeo. Questa Nota di aggiornamento, in particolare, è quindi densa del contenuto delle due manovre d'estate. Il documento, cioè, evidenzia come, in un contesto difficile in cui cominciavano a riscontrarsi tensioni sui mercati finanziari e sui debiti sovrani, per fronteggiare i possibili rischi derivanti da tale contrazione del PIL, il Governo abbia deciso di accelerare nell'attuazione dei due decreti-legge che hanno composto la manovra correttiva di finanza pubblica. Ricordo, infatti, che il Documento di economia e finanza aveva previsto un percorso di riduzione dell'indebitamento, volto a conseguire l'obiettivo di medio termine del pareggio di bilancio nel 2014, attraverso una manovra correttiva, però, da realizzarsi prevalentemente nell'ambito degli esercizi 2013 e 2014. La Nota in esame, pertanto, pone in risalto come, per fronteggiare i possibili rischi derivanti da tale contrazione del PIL e in un contesto nel quale cominciavano a riscontrarsi tutte queste tensioni, il Governo abbia anticipato, a luglio e ad agosto, le misure previste. Questo noi oggi registriamo, perché, mirando a raggiungere il pareggio di bilancio nel 2013, cioè un anno prima rispetto a quanto ipotizzato nel DEF, con una correzione netta cumulata pari

ad agosto, il debito pubblico può seguire un sentiero di ancor più rapida riduzione, nel senso che, pur confermando le stime già presenti nel DEF, registrerà, comunque, una diminuzione più marcata negli ultimi due anni, fino a raggiungere il 112,6 per cento in rapporto al PIL nel 2014. La peculiarità della situazione che questo documento descrive trasferisce quindi la Nota di aggiornamento all'interno di una discussione dal contenuto specifico. Nel nuovo contesto di*governance* economica, esso non è più un documento eventuale, da presentare nel caso di scostamenti rispetto agli obiettivi e alle previsioni inizialmente individuati, ma diventa un documento documento necessario, inserito a pieno titolo tra gli strumenti di programmazione individuati dall'articolo 8 della legge n. 196 del 2009. Nel caso odierno, però, la Nota registra essenzialmente gli effetti delle rilevanti correzioni già realizzate, pur non mancando elementi per avviare un dibattito su possibili ed ulteriori interventi da realizzare. La strada da perseguire è quindi - e ce lo siamo detti più volte - quella delle riforme. Certamente mantenere il livello di severità contabile fin qui raggiunto è è necessario, ma non bisogna sottovalutare gli effetti recessivi derivanti da una contrazione troppo forte della domanda interna. Quindi, ancora una volta, il consolidamento dei conti pubblici è necessario per conseguire gli obiettivi, progressivamente più ambiziosi, concordati con le istituzioni europee, ma occorre porre solide basi per una crescita duratura nel medio periodo: per fare questo, occorre accompagnare quel rigore a misure di stimolo alla crescita. Penso a quelle già attuate dal nostro Governo, a quelle introdotte dalla manovra estiva, che vanno a rafforzare la sostenibilità del sistema pensionistico, ad esempio, cioè il progressivo innalzamento dell'età pensionabile da 60 a 65 anni delle donne occupate nel settore privato, per allinearla con quella degli uomini nel 2026. di legare l'età pensionabile alle aspettative di vita dal 2013 o al posticipo delle finestre di uscita dal mondo del lavoro. Vorrei rispondere al senatore Morando, che stamane, proprio su questo tema, ci incalzava, ed incalzava l'Aula, ad avere più coraggio e a fare di più. Come non ricordare, senatore Morando (giro ovviamente questa mia riflessione ai colleghi dell'opposizione), che dell'opposizione), che l'eliminazione di quel cosiddetto scalone Maroni fu voluta proprio dal Governo Prodi, proprio quando l'attuale opposizione era maggioranza, quando il senatore Morando era Presidente della Commissione bilancio. Come si fa oggi a chiedere il contrario di ciò che è stato fatto qualche anno fa dal Governo che la maggioranza dell'epoca sosteneva? abbiamo provato a farlo, qualcuno lo ha disfatto, oggi riproviamo a farlo, perché noi continuiamo a portare avanti con responsabilità le misure che ci sono state raccomandate dall'ECOFIN a sostegno del piano di consolidamento che l'Italia si è impegnata ad attuare per correggere il disavanzo eccessivo. ad esempio, alle misure contro la disoccupazione, alla riforma del contratto collettivo, alla commisurazione tra aumenti salariali e di produttività o alla liberalizzazione dei servizi. Spero che la lettera firmata da Trichet e da Draghi abbia messo la parola fine ad inutili polemiche che danneggiano solo la credibilità del nostro Paese. Io penso sempre che, tra le riforme strutturali che vanno messe velocemente in cantiere, e che questo Governo ha messo velocemente in cantiere, ci sia prima tra tutte proprio quella fiscale. fiscale. Ha ragione il senatore Morando, quando stamattina ha ricordato l'aumento della pressione fiscale, in ordine soprattutto alla diminuzione di quel denominatore fondamentale che è la produzione del PIL.

e non allo scopo di contenere e ridurre la spesa pubblica o di migliorare la qualità dei servizi, ma solo per dare copertura a nuove spese. In questo, forse, sta tutta la differenza di visione tra questa maggioranza e quella che era la maggioranza dell'epoca. Per noi, quella riforma ha il compito di rivedere l'insieme del sistema dei trasferimenti, di intervenire sull'IRE, sull'IRES e sull'IRAP per per razionalizzare il sistema tributario, alleggerendo il gravame per i contribuenti, soprattutto per quelli più deboli - quelli che ha ricordato il senatore Giaretta - e spero che ciò si possa fare anche con il contributo dell'opposizione.

verso la capacità di rilanciare lo sviluppo del Paese, e questo Governo, dal primo giorno del suo insediamento, lo ha avuto sempre in mente e continua,

si è complicata gravemente a livello generale e si presenta oggi come crisi strutturale e profondissima: una crisi - per intenderci - di quelle che dureranno a lungo e di cui tutti conservano la memoria. In questa situazione, negli ultimi mesi, il Governo ha presentato in Parlamento tre manovre, l'ultima delle quali ha conosciuto cinque riscritture. Nel frattempo, dopo aver perduto l'occasione della discussione sul DEF, allorquando il ministro Tremonti ostentava una rappresentazione ottimistica della situazione italiana e ci assicurava che il Paese e i suoi conti erano assolutamente in linea con l'Europa, l'Italia è stata, tra tutti, il Paese più esposto e il Governo non ci ha mai detto perché. Perché siamo arrivati a questo punto in pieno agosto? Non è mai stata data al Paese e al Parlamento una spiegazione, una ragione del come sia stato possibile arrivare ad essere i più esposti, i più a rischio, in Europa e per l'Europa. Non l'ha fatto semplicemente perché è la situazione politica italiana ad essere nel cuore di questa crisi. Purtroppo non lo diciamo solo noi, che siamo l'opposizione politico-parlamentare: imprenditori italiani, per la prima volta, lo gridano a gran voce.

per i cittadini onesti che pagano le tasse, per i giovani che non hanno alcuna responsabilità per il debito accumulato, per le donne che hanno visto disatteso ogni impegno nei loro confronti relativo al *welfare* in cambio dell'aumento dell'età pensionabile, e mancanza di rispetto per il Parlamento. Già, perché noi qui oggi siamo chiamati con la Nota di aggiornamento, tra l'altro, a verificare le maggiori entrate dei provvedimenti che sono già stati assunti e che hanno disposto norme di contrasto all'evasione fiscale, come - ad esempio - quelle che riguardano la partecipazione dei Comuni all'accertamento tributario, la riduzione del segreto bancario, la revisione della disciplina relativa alle società di comodo e molto altro ancora. il Presidente del Consiglio sta chiamando la sua maggioranza a schierarsi tutta a favore di un nuovo condono fiscale ed edilizio, per fare cassa e - si dice - per la crescita, quando tutti sappiamo che il Governo non è mai stato capace neanche di esigere il ristorno dei condoni precedenti e Banca Italia ci ricorda che ogni anno si perde qualcosa come 120 miliardi con l'evasione fiscale. Ora, come possiamo stupirci della perdita di credibilità che ci caratterizza nel contesto internazionale? Dall'Europa arrivano messaggi sempre più preoccupati. Trichet, questa mattina, ha detto che abbiamo il tempo contato e che la gravità della situazione richiede decisioni chiare. Nella vicenda politica italiana prevale la palude, il rischio dell'avvitamento e del trascinamento, e questo perché il centrodestra mette i propri interessi, e non quelli del Paese, al primo posto. Per questo, solo per questo, vuole restare comunque a galla, vuole comunque governare fino all'ultimo giorno, a qualunque costo e a qualunque prezzo per il Paese. La disinvoltura con cui, in questi

da ultimo con l'introduzione del famigerato articolo 8 dell'ultima manovra finanziaria. Tuttavia, sia ben chiaro che, nonostante tutto questo, nonostante la nostra consapevolezza che questo Governo non è nelle condizioni di servire il suo Paese, noi continuiamo a badare al merito e ad avanzare proposte, perché sappiamo che comunque è questo - e non un altro - il momento di agire e ci assumiamo tutte le responsabilità che ci competono come forza di opposizione in questa difficile e tristissima situazione italiana. economia e finanza conferma le condizioni di anticipazione del pareggio di bilancio al 2013, esclusivamente però per effetto della piena realizzazione di tutta la manovra. Un primo serio problema in tal senso è rappresentato dall'aleatorietà delle variazioni previste sulle entrate per effetto della riduzione dei regimi di favore fiscale ed assistenziale, per la quale si prevedono maggiori entrate per circa 20 miliardi di La stroncatura della Corte dei conti, che giudica generici i contenuti della delega fiscale e incerta la copertura, è un primo atto, che ci dà conto del rischio che venga pregiudicata tutta la manovra e conseguentemente il previsto pareggio di bilancio. evidente che la previsione di effetti positivi per 20 miliardi di euro ha come fonte principale quella dei tagli all'assistenza, ovvero i tagli previsti nella delega, dove si fa testualmente riferimento all'abrogazione delle leggi attualmente vigente in materia vigente in materia di tributi, nonché in materia socio-assistenziale. Non è difficile immaginare che il Governo si appresti a cancellare la legge n. 328 del 2000 e con ciò a comunicarci quello che realmente intende fare per riformare l'assistenza - in un contesto di così grave crisi, di disastro occupazionale, di povertà crescente - ovvero tagliare i diritti delle persone più deboli e delle famiglie. evidente l'assoluta mancanza di coerenza tra la delega fiscale e assistenziale e la legislazione federalista già approvata. È certamente interessante però che il Governo, con il documento in esame, riconosca gli effetti recessivi della manovra adottata

possa produrre effetti non positivi - che è come dire: «effetti negativi» - sul tasso di crescita del prodotto, che secondo la Nota sarebbero tuttavia controbilanciati da ulteriori effetti positivi a seguito - così si dice - dell'attivazione di meccanismi «non keynesiani». Si ipotizza cioè che in presenza di un miglioramento e del risanamento della spesa migliorerebbero le aspettative degli operatori economici, migliorando in tale modo sia la propensione ad investire sia quella a consumare.

Il portato di queste politiche è già verificabile oggi nell'accrescimento dei divari che contraddistinguono il nostro Paese: quello tra le generazioni, quello tra uomini e donne e quello territoriale, tra Nord e Sud. Vorrei soffermarmi solo Il risultato della politica economica del Governo e delle manovre adottate è che si sono ulteriormente acuite le divaricazioni che interessano tutte le regioni del Sud. è maggiore la contrazione della spesa per le famiglie e dei consumi, è iniqua la ripartizione della riduzione di spesa, che investe di più le regioni del Sud,

effetti ingiusti delle manovre sono evidenti perché pagano i più deboli, pagano i più poveri, i giovani e le donne. Si è definitivamente rotto un modello di sviluppo e il mercato del lavoro vede al Sud un impatto negativo che è doppio rispetto al Nord: ci sono meno iscritti all'università, ci sono più laureati ma non lavorano e non studiano più, le giovani donne meridionali non sono più le più prolifiche, anzi, sono state superate dalle giovani del Nord.

e noi non dovremmo porci l'obiettivo di un grande programma per il lavoro dei giovani e delle donne? Il credito d'imposta per le assunzioni a tempo indeterminato nelle regioni meridionali ha avuto finalmente venerdì scorso il via libera della Commissione europea. Oggi dunque disponiamo di un nuovo strumento di sostegno alla creazione di nuova occupazione, automatico ed incentivato, che riscuote anche il gradimento delle imprese. Ora serve una strategia, che fin qui non è stata praticata, che indichi una nuova frontiera per lo sviluppo italiano, una ripartenza dal Sud verso il Mediterraneo e verso l'Europa. Questo è quello che ci chiedono i tanti giovani che manifesteranno sabato a Roma e anche tutti gli altri che sono troppo preoccupati per manifestare; questo è quello che una politica solamente seria dovrebbe fare. La maggioranza non lo vuole fare. Lo faremo certamente noi.

so che alcune cose che dirò sono già state poste all'attenzione di quest'Aula da chi è intervenuto prima di me, ma credo sia doveroso ribadire che dalla lettura di questa Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza non si possono trarre motivi di ottimismo per quanto riguarda il futuro del nostro Paese, la sua crescita e la sua capacità competitiva. Le prospettive di crescita per il medio termine sono quasi inesistenti ed il *mix* degli interventi messi in atto nelle due manovre estive non restituisce alcuna credibilità al nostro Paese. La pressione fiscale effettiva è destinata a crescere -come è stato ricordato stamane dal collega Lannutti - ben al di là delle ultimissime stime del Governo. In questo momento pare altamente improbabile che si possa giungere all'approvazione della delega fiscale entro il settembre 2012: occorrerebbe un Governo unito, coerente, credibile e, soprattutto, disposto, una volta tanto, ad occuparsi dei problemi dei cittadini piuttosto che delle beghe interne ai partiti di maggioranza. E così alla fine, guarda caso, sarà la clausola di salvaguardia ad assicurare il maggior gettito, il che vuol dire, in sostanza, che si opererà con tagli alle agevolazioni fiscali e assistenziali tuttora presenti nel nostro sistema. Quella delle infrastrutture dovrebbe essere la prima battaglia di un Paese che vuole crescere, e non certo attraverso colate di cemento o sabbia e ghiaia, ma innanzitutto attraverso una migliore definizione del quadro finanziario di riferimento, una più adeguata programmazione e individuazione delle opere, una più efficace suddivisione dei compiti tra i diversi livelli di governo, un vero monitoraggio sui tempi, sui costi delle opere e sull'effettivo soddisfacimento dei bisogni infrastrutturali. La mancanza di una disciplina finanziaria nei processi a monte ha portato alla necessità di un sistema di controllo delle erogazioni a valle; questo ha fatto sì che si è finito con l'ampliare ulteriormente la lista delle opere potenzialmente finanziabili. A distanza di quasi dieci anni dall'introduzione della legge obiettivo non si sono registrate accelerazioni nei tempi di realizzazione delle opere, né si è sciolto il nodo dei finanziamenti. E soltanto ora, nell'Allegato «Infrastrutture», si accenna ad una autocritica dello strumento. D'altronde, non era possibile fare altrimenti, considerato che nel frattempo è stato divulgato il VI Rapporto sull'attuazione della legge obiettivo redatto dal Servizio studi della Camera, in collaborazione con l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici. Dalla lettura di tale Rapporto, infatti, non sembrano ricavarsi elementi che ci permettano di giustificare un mutamento di giudizio sull'inadeguatezza, anche alla luce di una generalizzata e gravissima situazione di crisi economica, della politica del Governo in materia di infrastrutture. Ma non basta. Non si parla, infatti, nel primo paragrafo del documento dedicato alla legge obiettivo, del tema del centralismo che ha caratterizzato la stessa legge, massimizzando così gli sprechi. Infatti, provenendo le risorse per le infrastrutture dall'amministrazione centrale, l'obiettivo delle *lobbies* industriali e locali è sempre stato, in questi anni, quello di massimizzare i trasferimenti, non certo di garantirne l'efficienza. Attenzione: ad oggi, nel Programma di infrastrutture strategiche sono comprese 390 opere, a fronte di un primo elenco che ne conteneva 110, soltanto 21 delle quali erano considerate veramente strategiche. Ma quello che lascia davvero sconcertati - e che dovrebbe interessare anche l'Aula un po' disattenta - è che di queste opere, in 10 anni, ne sono state ultimate soltanto 30 e poco più del doppio sono quelle per cui hanno avuto inizio i lavori. Mancano ancora da reperire 217 miliardi di euro. È la relazione della Corte dei conti sul rendiconto 2011 che ci ricorda che si è rinunciato all'essenziale preminenza programmatoria dello Stato. In primo luogo - si legge è stato mancato l'obiettivo di fondo, cioè la selezione di un numero ridotto di interventi infrastrutturali ad alta priorità strategica. Sono, pertanto, divenuti prioritari progetti di opere di interesse soltanto locale, ovvero completamenti di interventi già in corso o, ancora, progetti di grande impatto di annuncio, ma privi dei necessari elementi di valutazione economico-finanziaria o di fattibilità. In alternativa, si sarebbero dovuti predisporre programmi diversi, dedicati a poche nuove infrastrutture realmente strategiche, ai più urgenti completamenti di opere in corso e ai principali colli di bottiglia non li cito perché sono noti - e forse anche un ultimo relativo alla manutenzione e alla messa in sicurezza del territorio e delle opere. Il modello seguito in Spagna dovrebbe farci riflettere, perché coniuga le due varianti fondamentali: finanziamento e programmazione. In Spagna si è proceduto attraverso una stringente opera di selezione ed il perseguimento di poche priorità nazionali, ma anche introducendo un innovativo meccanismo d'asta per contenere e allocare le spese compensative collegate alle opere. Nell'allegato viene poi prospettata una nuova strategia finalizzata a valorizzare e rafforzare l'offerta portuale nazionale. Non c'è bisogno che io mi trattenga su questo punto, sappiamo bene quale è la situazione: stiamo perdendo competitività giorno dopo giorno. Mi riferisco ai porti di Gioia Tauro e Taranto, che tra i porti di *transhipment* vivono il periodo peggiore. Nel porto calabrese oltre il 40 per cento della forza operativa del *terminal* è in cassa integrazione; il cliente più importante del porto - Maersk Line - da metà anno non porta più le sue navi in banchina. Un primo crollo c'è stato a luglio, e si teme che alla fine dell'anno si arrivi a registrare una flessione di *container* che dovrebbe essere oltre Credo che questi siano i dati che debbano interessare il Paese ed i senatori. A Taranto, Evergreen Line*,* operatore di Taiwan, ha deciso di spostare tre servizi sul porto del Pireo in Grecia. Come si pensa di ovviare allora a queste situazioni? L'allegato a noi non dà alcuna risposta, alcuna indicazione. Si prevede poi la definizione di*action plans* nell'offerta aeroportuale, ossia dei piani attuativi mirati in grado di adeguare l'intera rete aeroportuale alla crescita del traffico del prossimo ventennio. Ci si dimentica di affrontare, però, il problema dell'assetto del mercato, che fa sì che gran parte degli scali piccoli e medi italiani chiuda il bilancio stabilmente in passivo; che nel settore aeroportuale la liberalizzazione sia ancora parziale, a causa delle barriere all'entrata legate ai meccanismi di allocazione degli *slot* orari di decollo e atterraggio, e per la concessione di sussidi e norme di favore verso l'operatore dominante. Basti pensare alla situazione in cui versa l'aeroporto di Ciampino per capire quali potrebbero essere i problemi per l'aeroporto di Viterbo, di cui parla il documento al nostro esame. Se, come ha detto qualcuno, la crescita del Paese passa anche dai porti e dagli aeroporti, allora sappiamo bene che, allo stato dei fatti e vista l'assenza di misure del governo in tali ambiti, non cresceremo affatto. Si scopre leggendo questo documento che urge una riforma del sistema dei trasporti: quello relativo alla movimentazione delle merci e quello legato al trasporto pubblico. Operatori dei trasporti, amministratori e accademici hanno evidenziato un ridotto grado di interconnessione tra le reti di trasporto in Italia. L'assenza nel nostro Paese di una politica capace di fare sistema tra tutti gli operatori della logistica per accrescere la competitività del Paese fa sì che il comparto logistico sia in grande difficoltà, dovendo collegare una struttura produttiva frammentaria e dispersa sul territorio, utilizzando delle infrastrutture poco interconnesse e un comparto merci delle ferrovie in ripiegamento. Viviamo in un Paese in cui negli ultimi anni il settore del trasporto pubblico locale è stato interessato da logiche di contenimento dei costi e riduzione della spesa pubblica che, avulse da qualsiasi riflessione di contenimento selettivo, di rilancio del settore e miglioramento del servizio pubblico universale, sono senza alcun dubbio alla base delle gravi inefficienze e degli ostacoli che non assicurano al cittadino la garanzia del diritto alla mobilità. Nessuno di questi elementi viene considerato dal documento, mentre si parla della funzione strategica solo dei pedaggi stradali e ferroviari. Non è una scelta impopolare quella di far pagare il pedaggio sui tratti stradali che presentano caratteristiche autostradali: è una scelta sbagliata, soprattutto se non esistono, nel sistema viario territoriale, strade funzionali alternative, perché il pedaggio finisce per penalizzare migliaia di cittadini. Secondo il calcolo delle associazioni dei consumatori, l'introduzione del pedaggio sui raccordi autostradali costerebbe mediamente 600 euro annui ai lavoratori pendolari. Allora, che dire: è evidente che occorre un cambio di strategia che non avete cercato e voluto (mi riferisco al Governo). Con la vostra politica economica e finanziaria non avete portato il Paese da nessuna parte, ma solo alla stagnazione e all'immobilismo. Ma quello che è più grave è che, anche in prospettiva, sembra che non vogliate e non riusciate ad invertire la rotta. È questa l'Italia che voi volete? Non la vogliamo noi. Forse è meglio che vi fermiate e lasciate il passo.

Questo plasticamente dà l'idea di quello che sta avvenendo. Fatta questa premessa, considerazione sempre legata a questa riunione. In quella sede si parlava del futuro dei fondi di coesione, cioè la nuova programmazione dei fondi di coesione dopo il 2013.

del cosiddetto equilibrio macroeconomico, cioè alla capacità del Paese di essere a posto con determinate poste di bilancio (per quanto ci riguarda, ovviamente, il debito, il piano di rientro e quant'altro). Il rischio che il nostro Paese subisca una decurtazione forte di questi fondi dunque è abbastanza

Ebbene, trattandosi di un rapporto, si può agire sul denominatore, cioè sulla crescita, oppure sul numeratore, cioè abbattendo il debito.

Anche questo, probabilmente, ce lo dobbiamo dimenticare. Vengo quindi alla questione dei tagli lineari, spesso - giustamente - molto criticata.

gli incentivi possono teoricamente andare bene soltanto per attivare un percorso; nel momento in cui si mantiene l'incentivo, quell'azienda, quel mercato o quel settore rimane drogato dall'incentivo e di fatto non funziona come dovrebbe.

gli interventi finanziari offerti dal Governo e dalla sua maggioranza a fronte della più grave congiuntura economica dal dopoguerra ad oggi (nonostante il quadro prospettato dal Documento di economia e finanza aggiornato con l'odierno provvedimento e nonostante nonostante l'ormai superato decreto sviluppo e le due manovre finanziarie di luglio e di agosto), non sono riusciti a far vedere agli italiani la luce in fondo al tunnel della crisi. La responsabilità dell'attuale situazione non è certamente imputabile solo a fattori esogeni: l'indebolimento delle prospettive economiche mondiali e la crisi dei mercati internazionali, più volte evidenziati dal Governo nella Nota di aggiornamento al DEF 2011, non sono i soli fattori costitutivi della gravità del momento che gli italiani stanno vivendo. Molto è dipeso anche da fattori interni, riconducibili spesso a scelte sbagliate e confuse, adottate da questo Esecutivo e sostenute dalla sua maggioranza sin dall'inizio di questa legislatura; dalla incapacità di dare una risposta di prospettiva alla gravità della situazione che intervenisse sul rilancio della crescita e dello sviluppo;

che individuassero le misure da adottare non in interventi di maggiori entrate, attraverso l'aumento della pressione fiscale, bensì in doverosi e non più rinviabili interventi strutturali di riduzione della spesa pubblica, almeno di quella improduttiva. La legge di contabilità e finanza pubblica prevede che la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza indichi «...l'eventuale aggiornamento degli obiettivi programmatici (...) anche al fine di stabilire una diversa articolazione di tali obiettivi tra i sottosettori». La Nota in esame, invece, non propone una nuova articolazione degli obiettivi di indebitamento netto per sottosettore, anche se l'accelerazione del percorso di consolidamento potrebbe influire sulla ripartizione proposta lo scorso aprile.

Il tentativo non riuscito di risanare i conti pubblici - con un debito pubblico che ha superato i 1.911 miliardi di euro, una pressione fiscale che alla fine del 2013 potrebbe superare il 45 per cento, l'assenza di numerosi miliardi di euro per far quadrare i conti delle ancora insufficienti due manovre estive - vede nella Nota di aggiornamento in esame il provvisorio epilogo di questo deplorevole itinerario.

di fronte alla quasi impossibilità che il PIL del nostro Paese crescesse nel secondo semestre 2011 dello 0,7 per cento, avete messo, come gli struzzi, la testa nella sabbia. È stata necessaria una lettera della Banca centrale europea che commissariasse di fatto il nostro Paese, umiliando le istituzioni di Governo della Costituzione repubblicana, per obbligare il Governo Berlusconi ad anticipare al 13 agosto un Consiglio dei ministri già convocato per il 18 agosto che, adottando, a volte in modo sommario, alcuni provvedimenti richiesti dalla Banca centrale europea, di fatto rendesse spiegabile all'intera opinione pubblica europea, compresa quella contraria, il massiccio acquisto di titoli pubblici del nostro Paese da parte della Banca centrale europea, con lo scopo di ridurre lo *spread* fra i mitici *Bund* tedeschi e i nostri BTP, alleviando parzialmente la tensione sui mercati internazionali ed offrendo alla Banca centrale la giustificazione per quella scelta di politica monetaria europea con una sorta di affidabilità del nostro Paese asseverata dalle decisioni ferragostane. Il fato ha voluto che la crisi del Governo e della maggioranza che lo sostiene stia coincidendo e sia precipitata proprio in un momento di particolare crisi economica nella quale il nostro Paese è chiamato da subito ad adottare

bloccato dalla inadeguatezza di questa maggioranza, rischi di non vedere tutelati i propri cittadini adempiendo agli impegni assunti. Abbiamo dovuto attendere la pubblicazione della lettera della Banca centrale su un famoso quotidiano nazionale, solo pochi giorni fa, per leggervi cosa avessero scritto Trichet e Draghi al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia del nostro Paese. Infatti, alla richiesta degli italiani - non vedo la collega Bonfrisco che di questo ha parlato in parlato in precedenza - di conoscerne il contenuto era stata opposta una riservatezza di maniera, quasi una clausola di stile e di buona educazione, come se gli italiani non fossero sufficientemente interessati, ciascuno in prima persona, al contenuto di quella missiva, che poi - come ne abbiamo avuto conferma - li riguardava direttamente tutti e in prima persona. La Nota di aggiornamento del DEF prova a prendere finalmente atto del mutato quadro economico, evidenziando, rispetto alle previsioni dell'iniziale Documento, una forte diminuzione del *trend* di crescita dell'economia del nostro Paese di ben 2 punti percentuali nel periodo 2011-2014: circa 35 miliardi di euro nel quadriennio. Ma un dato è ancora più preoccupante: la nostra economia va e andrà sistematicamente peggio di quella degli altri Paesi europei. Ce lo dicono ancora una volta i vostri dati: ammettendo che per il 2011 il PIL italiano sia stimato crescere solo dello 0,7 per cento rispetto all'1,1 per cento indicato in precedenza, bisogna reperire, solo per questa voce, quasi 7 miliardi di euro di minore crescita. Una crescita ancora più modesta è attesa per gli anni 2012-2013, nei quali il PIL è stimato, rispettivamente, allo 0,6 per cento e allo 0,9 per cento. Ciò per non parlare del 2014, quando la crescita si assesterebbe intorno all'1,2 Ma le stime di crescita, così come enunciate nella Nota di aggiornamento, divergono da quelle formulate dal Fondo monetario internazionale, che invece indicano, per il nostro Paese, un andamento negativo in rapporto al resto dei Paesi maggiormente sviluppati. Ecco perché non è più rinviabile che il Governo chiarisca se, dato il vincolo del pareggio di bilancio che si vuole instaurare e che ci si è prefissati, il quadro previsivo formulato nella Nota tenga o meno conto di ulteriori nuovi interventi di politica economica volti a migliorare ulteriormente le aspettative, ad esempio rimodellando la spesa pubblica al fine di orientarla verso categorie di spesa con moltiplicatori più elevati. È l'ISTAT, non il Partito Democratico, a confermare che a settembre 2011 gli andamenti sfavorevoli già registrati nei mesi precedenti rivelano un ulteriore calo sia della fiducia dei settori produttivi sia di quella dei consumatori. Dal punto di vista della crescita economica, i nostri principali *competitors* internazionali durante la crisi hanno registrato una minor riduzione percentuale del PIL e ora, nella fase di ripresa economica, registrano tassi di crescita molto superiori al nostro: lo conferma la previsione di crescita del PIL italiano nel 2011 stimata dello 0,6 per cento rispetto all'1,6 per cento dell'area euro: i numeri parlano chiaro. i numeri parlano chiaro. Per avviare la ripresa è necessario affiancare alle strategie di risanamento di bilancio le riforme strutturali, idonee ad elevare il potenziale di crescita economica del nostro Paese. Non lo diciamo solo noi, a quanto pare, signor rappresentante del Governo. Nella classifica dei Paesi a più alta competitività,

se è vero che le cose vanno male dappertutto in tutti i Paesi avanzati, da noi vanno peggio che altrove. E la collegialità del Governo sembra se ne sia accorta soltanto ora, dopo la lettera della BCE. Che la situazione fosse complicata lo sapevamo tutti, compresi voi che sostenete questo Governo, già dall'ottobre del 2008: da allora, avete messo in campo interventi insufficienti e non all'altezza della sfida. Oggi l'urgenza è quella di abbattere le sacche di dispendiosa e inutile spesa pubblica, combattere gli sprechi, attuare, ora che finalmente lo avete approvato, dopo 3 anni che ve lo proponevamo, quel processo di *spending review*, nel rigoroso e costruttivo rispetto dei tempi previsti nel convertito decreto-legge n. 138 del 2011, offrendo al Paese il risultato atteso: grandi risparmi di scala, così come prefigurato dal compianto ministro Padoa-Schioppa, che tanto avete bistrattato. Ancora: sostenere la crescita economica; rilanciare la domanda interna nel breve e nel medio-lungo periodo; mettere in campo, infine, una politica di riforme vere che accresca la competitività del nostro Paese, facendo ripartire lo sviluppo e la crescita con misure strutturali.

Signora Presidente, rappresentante del Governo, colleghe e colleghi, l'evoluzione per molti versi frenetica dell'economia e della finanza mondiale mai come in questo momento richiede che la programmazione delle risorse risorse pubbliche debba essere via via adeguata e aggiornata al cambiamento delle prospettive di crescita del prodotto lordo, con le inevitabili conseguenze e i riflessi sulle principali poste finanziarie dei conti dello Stato. A tale compito assolve in modo puntuale questa Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza, presentato dal Governo lo scorso aprile, e appunto adeguato alle attuali prospettive, nel quadro dell'economia mondiale. mondiale. Rispetto agli obiettivi determinati lo scorso aprile, con le manovre citate, a seguito della forte pressione dei mercati finanziari internazionali che ha determinato un'evoluzione negativa dello *spread* per i titoli di Stato italiani rispetto a quelli tedeschi, si è ritenuto sostanzialmente di dover anticipare l'obiettivo del pareggio di bilancio dal 2014 al 2013. L'effetto di tali interventi è di duplice natura, perché, se da un lato produce conseguenze immediate sui conti pubblici, con il contenimento delle spese e il conseguimento di nuove entrate legate essenzialmente all'aumento dell'aliquota IVA dal 20 al 21 dall'altro provoca effetti restrittivi sull'economia, considerata la rilevanza della spesa pubblica rispetto al complesso del prodotto lordo nazionale (siamo al 50 Effetti restrittivi che si sommano alle prospettive di sviluppo mondiale già riviste in senso negativo da parte di tutti i principali istituti internazionali, con riflessi, anche questi inevitabili, sulle stime relative al nostro Paese.

della minore crescita derivi dagli effetti delle manovre fiscali e quanta invece dalle più sfavorevoli prospettive economiche generali; neppure il Documento attuale si avventura in tali previsioni, anche perché occorre riconoscere che entrano in gioco fattori di varia natura, legati alle aspettative dei soggetti economici sia interni sia esterni. Ad esempio, una stabilizzazione della finanza pubblica, tale da garantire i conti dello Stato contrastando l'attuale percezione di volatilità, può indurre nei soggetti privati una maggiore propensione agli investimenti una capacità del sistema Paese di attrarre risorse dall'estero, tale da favorire un'eventuale crescita dell'economia reale, anche senza stimoli diretti. Tali effetti, per quanto prevedibili, non sono esattamente quantificabili, ma possono collocarsi in un orizzonte di medio e lungo periodo, mentre le restrizioni, dovute sia ad un aumento del prelievo fiscale che a una riduzione della spesa pubblica, soprattutto quella per investimenti, sono tali da produrre effetti sull'economia più ravvicinati nel tempo. Resta indubbiamente il fatto la fase di indebolimento della crescita italiana si colloca in un quadro in cui tutte le economie avanzate sono costrette a veder ridimensionate le stime che finora si erano fatte in ordine alla ripresa economica, dopo una fase di recessione tra le più lunghe e profonde che il mondo occidentale abbia dovuto subire nell'ultimo secolo. Tutto ciò in quadro in cui, invece,

tali da costituire comunque un traino rispetto al prodotto lordo mondiale. Così, se l'area Euro fa segnare una previsione di crescita del PIL pari all'1,1 per cento

di modo che il complesso delle economie avanzate cresce mediamente di qui al 2014 ad una velocità pari a meno di un terzo di quella dei Paesi emergenti, guidati dall'economia cinese, i cui dati di crescita del PIL nel prossimo triennio sono superiori nelle stime attuali al 9 per cento. Mai come in momenti sovviene alla memoria l'antico detto liberista «nessun pasto è gratis», perché una crescita più stentata di quella che si poteva auspicare ha messo gli Stati, o meglio i loro debiti, di fronte alla tragica prospettiva della sostenibilità dei medesimi, con conseguenze che potrebbero essere di una gravita imprevedibile, perché, sempre per ricorrere al gergo economico, è già stato sparato l'ultimo colpo in canna

che l'Italia può uscire da una percezione di debolezza che, a mio avviso, va ben oltre i fondamentali della nostra economia e del sistema Paese. L'Italia è per molti versi un sistema atipico rispetto ad altre economie occidentali, in particolar modo per la presenza di piccole e medie imprese, oppure per l'elevata quantità

e la scarsa presenza di uno spirito nazionale giocano certamente la loro parte nella costruzione di un'immagine del Paese più negativa della realtà. Al ristabilimento di una percezione più corrispondente al vero devono saper contribuire, ognuna nel proprio ruolo, tutte le parti politiche e sociali, evitando quell'accanimento al «tanto peggio, tanto meglio», all'inspiegabile desiderio di autodistruzione che spesso colpisce il nostro sistema istituzionale, sociale, mediatico e di conseguenza l'opinione pubblica interna e internazionale. Ma tornando al DEF e alla relativa Nota di aggiornamento, coerentemente con il difficile quadro internazionale, esso prevede una riduzione delle aspettative di crescita per l'Italia, riducendo la stima del PIL

che non solo colloca l'Italia tra i Paesi con minor crescita in un'area, quella europea che, come si è visto, è già essa stessa svantaggiata rispetto alla prospettive dei Paesi emergenti e degli Stati Uniti, ma che pone serie conseguenze sui conti pubblici e sul benessere delle famiglie italiane nel medio termine, conseguenze che nell'immediato rischiano di essere aggravate dalla natura restrittiva delle manovre pur necessarie ad assicurare la stabilità dei conti pubblici e l'azzeramento del *deficit* entro il 2013. Se i dati della contabilità nazionale appaiono dunque in costante miglioramento, sulla base delle previsioni e delle legittime attese che conseguono alle severe manovre poste in atto tempestivamente e doverosamente dal Governo, anche sulla base delle sollecitazione dell'Unione europea, con la lettera richiamata dal collega Lusi - dobbiamo, a mio avviso, evitare di guardare a queste proiezioni come al diagramma - mi si passi il paragone - del malato che va sfebbrando, non perché la sua malattia evolva verso la guarigione ma piuttosto perché è indirizzata verso l'esito più infausto! Non pare più sufficiente, ridurre all'1,3 per cento l'aumento della spesa corrente rispetto al PIL nominale. Siamo ancora in un'ottica di manutenzione della funzione pubblica che non corrisponde alla gravità della dimensione necessaria alle riforme da porre in atto, soprattutto per quanto riguarda la presenza dello Stato nell'economia, che va ancora ben oltre i necessari compiti di regolazione e garanzia della parità di condizioni del sistema previdenziale, per quanto attiene alla capacità di far fronte a una miriade di funzioni nei confronti di una società sempre più sfaccettata e meno omologabile che non nel recente nel recente passato. Credo che siamo in un momento in cui la politica può ancora, con un sussulto di orgoglio e credendo nella legittimazione che le proviene da un sistema rappresentativo, prendere in mano le sorti del Paese. Se non lo facesse finirebbe per dare credito a coloro che auspicano l'avvento di soluzioni tecniche di una sostanziale espropriazione della sovranità popolare, di cui il Parlamento è espressione, soluzioni tecniche che in questo frangente sarebbero ascrivibili a un commissariamento del Paese per opera delle strutture internazionali e comunitarie. Avere il coraggio dell'autoriforma, superare le realtà consolidate e mai passate al vaglio critico del principio costi-benefici è la forza che questo Paese può e deve avere. Noi crediamo che non si possa concepire lo sviluppo mondiale nato dalle basi del capitalismo di matrice occidentale come una partita a somma zero, ma guardiamo anche ad una crescita di quei Paesi che sono sempre cresciuti, di quell'occidente che è sempre cresciuto e che ha un effetto traino anche per le seconde e le terze file.

in via preliminare condivido l'osservazione secondo la quale la Nota è divenuta una fotografia di provvedimenti già adottati. però, ricordato che essa, peraltro la prima presentata in attuazione delle nuove disposizioni sul semestre europeo, nasce col grave *handicap* di essere stata presentata dopo le due importanti e urgenti manovre estive e quindi, in definitiva, in circostanze del tutto eccezionali. Il tema maggiormente richiamato negli interventi che si sono svolti è quello della bassa crescita. Si tratta di un tema al centro dell'attenzione della maggioranza e del Governo. In proposito, va nuovamente ricordato che è in preparazione un ulteriore provvedimento in tal senso. Per quanto riguarda il tema della credibilità delle stime relative all'economia italiana, occorre lamentare che, al momento della loro elaborazione, esse erano in linea con la media delle stime elaborate dagli organismi internazionali e da altri centri di ricerca qualificati. Pertanto, esse appaiono plausibili. È chiaro che qualsiasi prospettiva di ripresa, anche per il nostro Paese, è da raccordare con un quadro congiunturale che sconti il miglioramento dello scenario macroeconomico internazionale entro cui il nostro Paese possa tornare a cogliere le opportunità di una nuova fase espansiva. In proposito, va ricordato che anche la Commissione europea, con la dichiarazione del portavoce della Direzione generale di economia e finanza, ha ritenuto la manovra varata dall'Italia congrua rispetto all'obiettivo del pareggio di bilancio. Per consentire la discesa del rapporto tra debito e prodotto interno lordo occorre *in primis* far crescere il denominatore con provvedimenti a sostegno della crescita, fra cui gli interventi in materia di infrastrutture, liberalizzazioni e privatizzazioni e in favore del Sud, indicati nella Nota di aggiornamento. In proposito, va anche ricordato che il Governo sta provvedendo ad una ricognizione del patrimonio pubblico a valori di mercato. Con riferimento alle osservazioni emerse nel dibattito in ordine all'acquisizione di ulteriori elementi utili di valutazione riguardo ai meccanismi di tipo non keynesiano, si rileva in primo luogo l'esigenza di utilizzare opportune cautele nell'utilizzo di modelli econometrici al fine della stima degli effetti macroeconomici della manovra. Le reazioni del settore privato al mutato contesto potrebbero non essere infatti pienamente colte dai modelli in uso. Effetti negativi meno marcati o positivi potrebbero infatti emergere anche nel breve periodo, nei casi in cui, per effetto della credibilità della manovra, si verificasse un abbassamento stabile ed immediato del tassi di interesse a lunga scadenza ovvero i consumatori rivedessero al rialzo i piani di consumo, riducendo il risparmio precauzionale a causa di effetti ricardiani. Quando alle osservazioni relative all'aggiornamento del quadro programmatico di finanza pubblica negli anni 2011-2014 in merito alla stima della pressione fiscale, devo ribadire la correttezza della scelta del Governo di non imputare, fino all'attuazione della delega in materia, delle somme derivanti dalla revisione delle

nel conto delle pubbliche amministrazioni, come già illustrato in sede di relazione. In tal senso, è possibile ipotizzare che gli eventuali risparmi conseguibili dal lato assistenziale e previdenziale serviranno a sostenere e a razionalizzare con compensazioni le situazioni familiari di maggiore bisogno, piuttosto che essere destinati alla riduzione del prelievo fiscale. In merito poi al rischio di una restrizione dell'accesso al finanziamento bancario da parte delle imprese e delle famiglie, dovuto all'incremento dei tassi di interesse, va detto che un effetto di spiazzamento sui mercati finanziari dettato dalla situazione di finanza pubblica è senz'altro da riconoscere. Non bisogna tuttavia trascurare il fatto che la sostenibilità del debito costituisce un problema dell'intera economia nazionale e non solo della pubblica amministrazione, dovendosi raccordare anche con l'andamento più generale dell'economia e con le prospettive di competitività del sistema Paese. Un'ulteriore osservazione attiene al quadro delle azioni e degli interventi correttivi delineati nella Nota. Essa non sconta chiaramente gli indirizzi che pure sono oggi allo studio e che dovranno formare apposito oggetto di decisione legislativa circa l'eventuale ricorso ad operazioni di finanza straordinaria volte alla riduzione dello*stock* del debito pubblico, con connessa riduzione del carico della spesa per interessi, che oggi grava annualmente sulle spese pubbliche, a partire da interventi da adottarsi sul versante della cessione e/o valorizzazione dell'ingente patrimonio pubblico. L'opzione può essere considerata - come ho già detto nella relazione non solo per il diretto impatto a beneficio della sostenibilità a medio termine del debito, ma anche, se non sopratutto, per gli effetti che avrebbe direttamente ed indirettamente sulla gestione e sostenibilità della spesa corrente. Mi sia consentita poi una ultima riflessione. La sostenibilità del debito è entrata in crisi negli ultimi mesi non già solo per la dimensione in sé stessa del suo ammontare, quanto sopratutto per il drastico rallentamento delle prospettive di crescita economica del Paese. Occorre pertanto agire in maniera il più efficace possibile nel ricollocare il Paese su un sentiero di crescita stabile e duratura, da cui deriverebbe un rinnovato vigore del rapporto debito/PIL, facendo in tal modo coincidere l'azione di risanamento della finanza pubblica con una ripresa delle aspettative, che avrebbe un effetti immediato sulla riduzione dello *spread* dei titoli italiani rispetto a quelli tedeschi. Occorre dunque procedere nel senso della rapida implementazione con decreti aggiuntivi delle 39 misure di sviluppo adottate dal Governo negli ultimi mesi.

di un voto di particolarissimo rilievo politico ed è significativo che, tra i voti mancati al Governo, ci sia anche quello del Ministro dell'economia. debbo mettere in relazione la discussione che stiamo facendo sulla Nota di aggiornamento con il contenuto del consuntivo bocciato alla Camera.

perchè noi si possa valutare come i due avvenimenti si intreccino fra di loro e si possa, quindi, prendere anche le posizioni politiche necessarie. Le chiedo, inoltre, anche a nome del Partito Democratico,

Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, il presidente Zanda ha avanzato con molto garbo, ma con altrettanta puntualità, la richiesta di sospendere i lavori in atto.

Ritengo che ci siano valutazioni di ordine certamente politico da fare. Il Governo non ha

il Tesoro italiano dovrà collocare quantità significative di titoli sui mercati. Noi ci presentiamo a quell'appuntamento non avendo approvato il rendiconto, con un Ministro dell'economia che risultava in missione durante la votazione sul rendiconto, con dei provvedimenti sulla crescita che vengono rinviati di giorno in giorno e, a questo punto, non si sa esattamente quando saranno approvati.

quando vedono che non siamo in grado di approvare addirittura il rendiconto? Cosa possono pensare quando la maggioranza arriva a 290 voti su un provvedimento come il rendiconto? Francamente, credo che la sospensione chiesta dal senatore Zanda in questo momento sia necessaria, anche perché dobbiamo capire su che basi, ora, ragioniamo per il futuro. Allo stato attuale delle cose non è nemmeno chiaro quali possano essere le soluzioni tecniche da dare ad un problema che

Presidente, credo che si debbano fare due osservazioni. quello che è accaduto alla Camera ha un rilievo politico indiscutibile ed è legittimo che l'opposizione ponga il problema. È altrettanto vero, però, che accanto a questa questione, ineludibile dal punto di vista politico, c'è una questione un po' diversa rispetto al dibattito che stiamo svolgendo. Noi, infatti, stiamo per approvare un documento che è stato già approvato dalla Camera dei deputati e che responsabilità istituzionale vuole

Capisco che anche questo fa parte di una certa impostazione; io però sto cercando di fare una riflessione che mi sembra ovvia, senatore Morando, perché prima o poi, al di là delle comunicazioni del Governo e comunque vada la situazione politica, lei sarà il primo ad avvertire, per senso di responsabilità, l'esigenza di approvare

ha provveduto ad aggiornare le previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica unitamente agli obiettivi programmatici del DEF. In secondo luogo, ha fornito le indicazioni sul bilancio pubblico in prossimità della presentazione in terzo luogo, ha dato conto delle raccomandazioni approvate dal Consiglio dell'Unione europea; infine, ha riferito i contenuti e le sanzioni previste dal Patto di stabilità interno nonché i contenuti del Patto di convergenza. Riguardo alle stime presentate nella Nota di aggiornamento, si evidenzia una revisione delle prospettive di crescita dell'economia rispetto al DEF, per effetto sia del rallentamento dell'economia mondiale sia dei conseguenti riflessi sulla situazione interna.

Riguardo alla finanza pubblica, nel Documento di economia e finanza di aprile l'Italia si era impegnata a raggiungere l'obiettivo di medio termine del pareggio di bilancio entro il 2014. Tale pareggio doveva avvenire tramite la realizzazione di una manovra fiscale pari a circa 2,3 punti percentuali rispetto al PIL nel periodo 2013-2014, equivalente a un aggiustamento del saldo strutturale

Abbiate la compiacenza di far ribadire al Governo alcuni concetti che è necessario che il Parlamento sappia. Le valutazioni politiche le faremo successivamente. A metà agosto, dicevo, con il riemergere delle tensioni sui mercati finanziari e l'ampliamento dei differenziali di rendimento sui titoli del debito pubblico, il Governo ha varato un intervento fiscale aggiuntivo che ha incrementato la correzione complessiva, portandola a 59,8 miliardi in termini netti cumulati, pari a circa il 3,5 per cento del prodotto interno lordo. Quest'ultimo provvedimento ha consentito di realizzare il pareggio di bilancio - che non è poca cosa - delle pubbliche amministrazioni già nel 2013, anticipando di un anno quanto concordato in Europa e indicato dall'Italia nel DEF. Nel 2014, il Nel 2014, il saldo del conto economico delle pubbliche amministrazioni è previsto raggiungere un avanzo dello 0,2 per i conti dello Stato sono stati messi in ordine. La manovra fiscale consente altresì di ricostruire un ampio avanzo primario, pari al 5,7 per cento del PIL nel 2014, permettendo al debito di collocarsi in un sentiero stabile di discesa a partire dal 2012. Il debito pubblico in rapporto al PIL, pur seguendo il profilo discendente stimato nel DEF, presenta una riduzione più marcata

si tratta di un aggiustamento significativo. Devo ricordare che la Commissione europea, con una dichiarazione del portavoce della Direzione generale di economia e finanza, ha ritenuto la manovra varata dall'Italia congrua ed apprezzata, sottolineando che la piena applicazione delle misure approvate dal Governo consentirà il raggiungimento del pareggio di bilancio nel 2013, nonché la ricostituzione di un ampio avanzo primario idoneo a garantire

Mi auguro quindi che, in un momento così particolare della vita dell'Italia, anche sulla crescita ci sia univocità

ci ha spiegato che i conti sono in ordine. *(Applausi dal Gruppo PdL)*. A nome dell'Aula del Senato, vorremmo spiegargli che i conti non ci sono, perché è stato bocciato dall'altro ramo del Parlamento il Rendiconto dello Stato. Quindi, se lei avesse accettato quello che il Presidente le ha proposto, cioè di pronunciarsi sulle proposte di risoluzione, senza farci la sua relazione come se niente fosse (se lei mi consente), ci avrebbe permesso di guadagnare qualche minuto, e anche lei si sarebbe preso qualche applauso di meno, che non erano del tutto applausi di consenso - come forse comprende - dall'Aula. *(Applausi dal Gruppo LNP)*. Ringrazio i colleghi della Lega anche per questo incoraggiamento, che prendo ben volentieri. Vorrei chiedere al Presidente di sollecitare anche gli Uffici al fine di metterci nelle condizioni di valutare questo precedente, perché è evidente a tutti che ciò che è avvenuto alla Camera dei deputati non è solo - come si è detto - una battuta d'arresto politica (cosa evidente), ma è un fatto che ha delle implicazioni

per votare sull'aggiornamento del DEF. È per questo che, anche a nome dei colleghi del mio Gruppo, vorrei chiedere che la riflessione di questa ora di tempo, Presidente, sia accompagnata da una valutazione tecnica degli Uffici che dovranno analizzare questo precedente per evitare che si trovi una scappatoia politica ad una terribile botta politica, ma anche per le implicazioni

Presidente, intervengo nuovamente sull'ordine dei lavori. Non vedo nei banchi del Governo il Ministro dell'economia, del quale avevamo chiesto la presenza, questo è uno dei fattori che mi induce in qualche modo a denunciare un'evidente sottovalutazione da parte del Governo di un problema che si è aperto con la bocciatura alla Camera del rendiconto. lei sa io nutro per la sua persona, che in questo momento avrei immaginato naturale che l'Aula del Senato venisse presieduta dal Presidente del Senato, che evidentemente sarà impegnato in altre faccende, così come avrei immaginato naturale la presenza del Presidente del Consiglio. Ciò non accade per - ripeto - un'evidente sottovalutazione della gravità della situazione. Ma io adesso sono qui a chiederle formalmente, signor Presidente, che questa nostra discussione venga interrotta e che, alla ripresa, domani mattina, il Ministro dell'economia venga a spiegare al Senato come intende sciogliere la questione evidente che nasce, anche ai fini dell'approvazione della Nota di aggiornamento che noi abbiamo appena adesso iniziato a discutere,

che noi dovremmo approvare, e un presupposto che nella prassi parlamentare del nostro Paese è stato sempre considerato scontato. Ed è per questa abituale e continua approvazione del rendiconto che i due documenti vengono discussi contemporaneamente. Infatti, non era mai accaduto in Parlamento, esclusa una volta

questa concomitanza tra i due provvedimenti venisse in qualche modo messa in discussione dalla bocciatura del rendiconto da parte del ramo del Parlamento diverso da quello che stava discutendo la Nota di aggiornamento. Signor Presidente, questa vicenda ha degli effetti politici e costituzionali molto rilevanti. Lei certamente conosce, signor Presidente, un costituzionalista importante, il professor Pitruzzella, importante anche perché è un consulente della Presidenza del Senato, alla quale lei fa onore con la sua presenza. Mi permetto di leggerle come il professor Pitruzzella ha illustrato il caso che noi ci troviamo adesso ad esaminare: «La legge di approvazione del rendiconto consuntivo è senz'altro un legge priva di contenuti normativi. Con questo atto il Parlamento esercita un controllo sul documento contabile presentato dal Governo in cui sono riepilogati i dati relativi all'esercizio trascorso. Il Parlamento non può che prendere atto dei risultati presentati. Certo, non può modificare ciò che è già compiuto e,» alla sua attenzione, signor Presidente - «se il Parlamento votasse contro il disegno di legge, la conseguenza politica non potrebbe che essere la crisi di Governo». Questo dice la dottrina costituzionale del nostro Paese. E noi affrontiamo questa fase nella distrazione generale del Governo. Il Ministro dell'economia, richiesto dall'opposizione di essere presente in Aula, non viene. Il Presidente del Consiglio si è lanciato in una dichiarazione stupefacente, in cui afferma che si tratta di un disguido tecnico a cui verrà messo riparo. Un disguido tecnico, signor Presidente? Ma ci rendiamo conto di ciò di cui stiamo parlando? Io le chiedo formalmente, e lo faccio a nome del Gruppo del Partito Democratico, di chiedere formalmente al Ministro dell'economia di essere qui in Aula domani mattina. E le chiedo anche di interrompere questa discussione perché, francamente, noi abbiamo già subito sufficiente discredito, per non passare dal discredito al ridicolo. la discussione non può continuare. La prego di prendere atto di una situazione evidente e di disporre di conseguenza. E la ringrazio, perché sono certo che lei ne terrà conto. Signor Presidente, oltre alle considerazioni che il collega Zanda ha fatto in precedenza, e che io non ripeto, noi non possiamo, stasera, esaminare la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, perché manca il presupposto, cioè un bilancio dello Stato che sia asseverato dall'approvazione del rendiconto generale. Questo risulta, nella sostanza e nella forma, bocciato dalla Camera, perché la bocciatura dell'articolo 1 significa La Camera ha sospeso i suoi lavori convocando la Giunta per il Regolamento e la Conferenza dei Capigruppo per domani, per comprendere come procedere. Noi non siamo scollegati da questo procedimento. Non possiamo approvare qui una Nota di aggiornamento, quando poi alla Camera fanno qualcosa di diverso, o viceversa. Al di là delle considerazioni di carattere politico, che mi riservo di fare in conclusione del mio intervento dal punto di vista squisitamente procedurale, noi non possiamo più andare avanti fino a quando non sapremo ciò che accadrà in ordine a questo fatto gravissimo, inedito e, mi dispiace doverlo dire, surreale, che certifica uno stato di sciatteria che è ancora peggio della difficoltà politica: è proprio la strafottenza rispetto a doveri che sono fondamentali e che riguardano la certezza dei rapporti finanziari tra lo Stato, il sistema delle autonomie, i cittadini e l'Unione europea. Guardate, io mi auguro che dietro questa vicenda vi sia un malessere di carattere politico, perché, se non fosse così, sarebbe ancora più grave. La circostanza che il Ministro dell'economia non partecipi al voto, che non si sappia chi partecipa e chi non partecipa, che manchino i voti della maggioranza e che l'atto venga

assoluta non credibilità all'estero in un momento particolare. Credo pertanto che bisognerebbe recuperare un minimo di senso del decoro e del rispetto delle istituzioni che tutti noi rappresentiamo.

necessariamente e doverosamente la sospensione dell'esame del provvedimento e il rinvio di ogni deliberazione. Le spiego, signor Presidente, e lo dico anche ai colleghi dell'Aula.

Il primo è di sostanza, e riguarda il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, che al primo comma, in maniera molto chiara, senza bisogno di scomodare i costituzionalisti, dice che «le Camere» (cioè tutti e due i rami del Parlamento) «approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo». signor Presidente, noi siamo stati chiamati, sotto i riflettori di tutta Italia e di tutta Europa, l'11 agosto dal Ministro dell'economia che doveva

qui ancora stentiamo a rispettare quelli che sono i principi sacri, chiariti nella nostra Costituzione in maniera indelebile. Detto questo, signor Sottosegretario, non è casuale che la legge di contabilità, che è stata salutata da questo Parlamento come una riforma epocale, stabilisca un diverso ordine cronologico e temporale per i due atti: il rendiconto generale dello Stato, che va presentato dal Governo al Parlamento entro giugno, e poi ‑ e soltanto poi la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, che va presentata dal Governo al Parlamento entro il 15 settembre. È evidente che in questo filo logico e temporale c'è la necessità che i due provvedimenti siano strettamente connessi. Noi pertanto contestiamo fortemente l'affermazione fatta da alcuni colleghi della maggioranza, secondo cui i due provvedimenti non sono tra di loro collegati. Questo è un falso storico,

del documento - sottolineo, aprendo una parentesi, che tutta la Nota di aggiornamento del DEF incorpora i contenuti delle due manovre

la correzione apportata alla spesa dei sottosettori delle amministrazioni centrali e locali per l'intero periodo di previsione, riflette la composizione percentuale della spesa primaria delle amministrazioni pubbliche nel 2010 (ultimo anno di consuntivo)». Quindi, il legame forte, consequenziale, temporale e anche di contenuti tra i due documenti documenti è evidente, e non lo diciamo noi dai banchi dell'opposizione, ma lo scrive il Governo accompagnando la Nota. Ma vi è di più, signor Presidente. Noi riteniamo che non sia assolutamente possibile proseguire una discussione e soprattutto procedere a una votazione del provvedimento, perché stiamo votando votando non tanto un aggiornamento di previsioni, bensì un aggiornamento di previsioni su un conto consuntivo che non esiste, in quanto non è stato approvato dal Parlamento, perché l'articolo 1 è quello portante di tutto il provvedimento. Aggiungo, signor Presidente, per completezza che, come voi tutti ricordate, nel decreto approvato ad agosto un capitolo importante, incorporato poi nella Nota di aggiornamento del DEF, prevedeva espressamente una riduzione delle spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascuno Ministero, ridotte dell'1 per cento per ciascun anno, rispetto alle spese risultanti dal bilancio consuntivo relativo all'anno 2010.

Sulle manovre economiche, sulle fiducie chieste a ripetizione, di mortificazioni questo Parlamento ne ha avute abbastanza rispetto a un senso di responsabilità delle opposizioni. Ricordo la nostra responsabile presenza ai lavori sull'ultima manovra economica che, presentata come urgente, è stata modificata cinque volte di seguito nel giro di poche settimane.

il rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato e i rendiconti di tutte le altre amministrazioni periferiche sono approvati nelle risultanze

nel corso della discussione di questa mattina ho avuto modo di esprimere le mie valutazioni sulla Nota di aggiornamento del DEF e mi sono riferito in modo esplicito alla tavola 7a, che ha come titolo: «Conto della pubblica amministrazione a legislazione vigente». Da questi dati ufficiali, che il Governo ha presentato in Parlamento, ho tratto le mie considerazioni, cioè che la manovra di agosto

signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo e onorevoli senatori, come è già stato detto, non è un caso che la sequenza cronologica di questi documenti sia fissata secondo buon senso: entro giugno si approva il rendiconto, entro il 15 settembre si fa la Nota di aggiornamento del DEF e poi si approva la legge di stabilità per l'anno successivo. Si tratta di un dato incontrovertibile.

e agli anni dal 2011 al 2014, con i numeri preventivi, che incorporano la legislazione vigente. In questo momento la tavola ha

non è stata bocciata: è stato bocciato l'articolo 1 della stessa. *(Commenti dal Gruppo PD)*. Fermo restando che tutto il mio intervento ovviamente niente ha a che fare con

preminente rispetto al contesto legislativo nel suo complesso) è costruito con l'indicazione dei saldi. Questo rendiconto, invece, è costruito nel modo esattamente contrario, in i rendiconti delle Amministrazioni e delle Aziende autonome per l'esercizio 2010 sono approvati nelle risultanze di cui ai seguenti articoli». è il primo articolo che fa riferimento a tutti gli altri. Ove mai si approvassero tutti gli altri articoli, ben le risultanze saranno state perfettamente approvate.

non è stato né bocciato né approvato, ma è in discussione all'altro ramo del Parlamento. Ove si voglia semplicemente questioni che hanno riguardato questa vicenda (sempre in maniera analoga perché il caso preciso è inedito), bisognerebbe ricordare alcuni piccoli passi che rapidamente, signor Presidente, colleghi, vado Voglio ricordare, innanzitutto, che il rendiconto generale dello Stato per l'anno 2010 è stato approvato già in prima lettura da questo ramo del Parlamento con l'Atto Senato n. 2803, e ribadisco che non vi sono implicazioni di carattere formale che precludono il seguito della discussione della Nota di aggiornamento. La Nota di aggiornamento, infatti - quella di cui discutiamo - è disciplinata dall'articolo 10-*bis* della legge n. 196 del 2009. Questa norma si inquadra in quel contesto nel ciclo di programmazione e fa seguito all'approvazione del Documento di economia e finanza, che - come è noto - è già stato esaminato dal Parlamento con l'approvazione delle risoluzioni nel maggio scorso, quindi in assenza dei disegni di legge di rendiconto e di assestamento. Ribadisco: quelle risoluzioni sono state approvate in assenza del rendiconto, e avevano la stessa identica natura formale di questa. Andiamo avanti. La Nota in esame, infatti, aggiorna per gli anni 2012 e 2014 gli obiettivi di finanza pubblica stabiliti nel Documento di aprile essendo i saldi in essa contenuti essenziali ai fini della presentazione della prossima legge di stabilità.

riferendo non a questo che stiamo esaminando, ma a quello del quale questo è prodromico). Ebbene, quel disegno di legge - adesso di stabilità, prima legge finanziaria - è stato spesso presentato in Parlamento

presentata la legge finanziaria il 1° ottobre, il rendiconto e l'assestamento furono approvati il 30 ottobre. Ho citato questi due esempi, perché si trattava di due anni di seguito, 2007 e 2008.

e disegno di legge di assestamento c'è un solo nesso: quello che riguarda i criteri di copertura della legge di stabilità. Ma ovviamente tale questione - come è facilmente comprensibile - in niente afferisce al rendiconto dello Stato: bisogna stabilire le modalità di copertura di una legge che stabilisce per il futuro (il rendiconto - com'è noto - è una legge che afferisce al passato). Il disegno di legge finanziaria, presentato in taluni casi prima dell'approvazione definitiva dell'assestamento, ha

dal disegno di legge di assestamento non ancora approvato. Attenzione: sto parlando dell'assestamento; il rendiconto - ribadisco - non ha nessun nesso di attinenza con ciò di cui stiamo per discutere ed eventualmente approvare.

di contabilità) - i Regolamenti parlamentari non pongono nessun nesso di carattere procedurale tra assestamento e rendiconto,

di ripetermi - di approvazione definitiva di uno dei disegni di legge e di modifica dell'altro, con conseguente *iter* parlamentare. Dunque, l'autonomia è perfetta, non solo tra Nota di aggiornamento al DEF, di cui ci stiamo occupando, e provvedimenti di legge importanti, quali la legge di stabilità, ma addirittura vi è un nesso di distinzione evidente tra le due leggi le due leggi che normalmente vengono presentate insieme: rendiconto e assestamento. Signor Presidente, mi pare di aver illustrato le ragioni per cui il nostro Gruppo si oppone nostro Gruppo si oppone alla richiesta di sospensiva; comprende, ma naturalmente non condivide affatto, le ragioni politiche che portano i colleghi ad affermare la loro istanza, ma ritiene che il Parlamento debba procedere oltre per continuare l'*iter* del documento. Questo - dico ai colleghi di opposizione - renderebbe, anche agli occhi dei consessi internazionali, il pieno esercizio delle nostre facoltà. Siccome anche i colleghi ovviamente ci tengono tanto, sono certo certo che anche in questo caso pure loro rinunceranno, per fare in modo che si vada avanti speditamente. Signor Presidente, la Camera dei deputati, dopo la votazione sull'articolo 1 del rendiconto 2010, ha sospeso i suoi lavori e sta valutando quali siano le conseguenze politiche e anche tecnico-formali di questo voto.

questo punto. Deciderà la Camera quali siano le conseguenze da trarre da quel voto. è approvato il rendiconto. C'è un articolo che dice: è approvato il rendiconto; la Camera dei deputati vota e non lo approva: secondo me, vuol dire che il rendiconto è bocciato. In ogni caso non voglio insistere; faccio solo una previsione: secondo me, questa sarà la decisione che prenderà la Camera dei deputati e, se le conseguenze politiche che il Governo a mio avviso dovrebbe tirare da quel voto non saranno tirate, il Governo verrà al Senato ripresentando il rendiconto così com'era. Questa è la mia previsione proprio perché, secondo me, la Camera deciderà esattamente nel senso di considerare quel voto come risolutivo: la Camera ha bocciato il rendiconto dello Stato. Ma qui non ci occupiamo di fare previsioni su quello che deciderà la Camera. Una cosa è sicura: c'è stato un voto che potrebbe seriamente mettere in discussione l'approvazione del rendiconto 2010. Noi stiamo discutendo la Nota di aggiornamento del DEF - signor Presidente, lei può controllare - contiene la tavola 7a. Tale tavola è il Documento di economia e finanza, perché contiene il conto della pubblica amministrazione a legislazione vigente. In quella tabella voi leggete - basta che la prendiate - la colonna 2010 in cui sono fissati i dati del consuntivo 2010, quelli contenuti nel disegno di legge che la Camera ha appena respinto e sul quale in ogni caso oggi abbiamo la certezza che il procedimento di approvazione ha subìto un arresto assai serio (vedremo domani mattina quali saranno le decisioni della Camera). Ora, signor Presidente, l'argomento è presto sviluppato; è perfettamente vero quello che ha detto il presidente Azzollini: noi abbiamo spesso - non sempre, naturalmente - discusso e votato il DEF nella relativa risoluzione (allora si chiamava DPEF, ma la sostanza è la stessa) e la relativa Nota di aggiornamento, prima di votare il consuntivo. Se noi dovessimo appurare questo, tra di noi non ci sarebbe alcuna ragione del contendere, ma, signor Presidente, le faccio notare un'evidenza, e cioè che la scansione temporale delle votazioni è sempre stata fondata sul presupposto

è la 7a, ma, in ogni caso, la tabella di tutti i DPEF e di tutte le Decisioni di finanza pubblica -contenente il quadro di finanza pubblica a legislazione vigente sarebbe stata destituita di fondamento.

abbiamo un rovesciamento totale del senso del presupposto. Noi adesso siamo sicuri che il rendiconto non è stato approvato, perché il voto della Camera è su questo punto esplicito, tant'è vero che secondo me dovremmo rideliberare, se il Governo non prenderà atto della situazione, su quel punto. E noi cosa chiediamo? Non chiediamo di non deliberare, in assenza di delibera della Camera sul rendiconto e sulla Nota di aggiornamento. Chiediamo di farlo domani mattina sulla base di un argomento che è elementare: dica il Ministro dell'economia, venendo al Senato, come intende ridare legittimazione e forza alla Nota di aggiornamento affrontando il problema che è stato creato dal voto della Camera. Non chiediamo niente di più di questo, e negarlo, francamente - fatevelo dire, colleghi della maggioranza - è, secondo me, assurdo, anche dal punto di vista dei vostri interessi.

Ma io presuppongo che non vogliate assumere questo orientamento e che quindi vogliate adottare una strategia di fuoriuscita, salvando il Governo dal voto che la Camera ha espresso. Se volete adottare questa strategia di fuoriuscita dovete farlo domani mattina sulla base di un disegno che abbia un minimo di coerenza, non pretendendo adesso di non fare un aggiornamento del dibattito che è nelle cose si debba fare, visto che la Camera sta sospendendo i suoi lavori in attesa di decidere come come trattare le conseguenze del voto che si è determinato. Ecco perché è perfettamente coerente non una richiesta di non votare fino a che non abbiamo approvato il rendiconto (perché nessuno di noi ha avanzato questa proposta), come abbiamo proposto - domani mattina sulla base di una comunicazione del Governo, che ci dovrebbe dire, nell'interesse del Paese,

in presenza di una crisi di fiducia che riguarda l'euro e riguarda la stabilità del nostro Paese, la solvibilità e la sostenibilità del debito pubblico italiano, abbiamo da introdurre il pareggio di bilancio strutturale nella Costituzione, non abbiamo nemmeno davvero seriamente cominciato quell'*iter* (ecco cosa spiega la differenza rispetto alla Spagna), alla Spagna), nel mentre, sul rendiconto abbiamo un voto della Camera che è quello che si è appena determinato. Ma volete prendervi il tempo per fare una valutazione e definire, nell'interesse del Paese, quale sia la strategia di fuoriuscita da questa situazione, quella, che voi, (quella che noi riteniamo utile l'abbiamo già detta cinquanta volte) ritenete utile per affrontare la situazione? Nell'interesse di tutti, secondo me questa sera dovremmo sospendere la discussione, essendo per noi pacifico che domani mattina si decide dopo che il Governo è venuto a spiegarci

se non avessi ascoltato le inarrivabili, in termini di scienza e di esperienza, espressioni del senatore Azzollini.

è stato respinto un articolo di tre righe che stabilisce: «Il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato e i rendiconti delle Amministrazioni e delle Aziende autonome per l'esercizio 2010 sono approvati

già altre volte è stato approvato il DPEF, o il DEF, senza che fosse stato approvato il rendiconto.

la Nota di aggiornamento in pendenza di questa gravissima crisi politica ed istituzionale. Forse il collega Azzollini pensa di usare la sua scienza per prenderci in giro.

Presidente, vorrei esprimere l'opinione del Gruppo di Coesione Nazionale-Io Sud-Forza del Sud

C'è un doppio problema: ce n'è uno politico, ma c'è anche un problema tecnico-procedurale. che definisco le sofisticate argomentazioni del presidente Azzollini - ovviamente non è convinto lui stesso di ciò che ci ha detto non possono convincerci. Se la Camera, a cui è stata affidata l'approvazione di un rendiconto che il Senato aveva già approvato,

Basta che lei legga, senatore Asciutti, il Regolamento anche quello della Camera. La prego di studiare ogni tanto! Il mondo va avanti, non è più fermo

ritengo che sia importante la sospensione, signor Presidente, per avere un quadro chiaro della procedura. Politicamente faremo tutti gli approfondimenti necessari, ma vogliamo evitare di sbagliare nelle tecniche di approvazione di un provvedimento legislativo.

Ho detto prima della sospensione che qui in Aula stiamo discutendo un documento diverso da quello in discussione alla Camera dei deputati. Mi sembra che la puntuale illustrazione del senatore Azzollini,

e quindi, a parte le offese a Bitonto e ad altre città fatte del senatore Rutelli, per le quali chiediamo noi scusa ai cittadini di quelle città, a nome del Senato, credo che la discussione politica sia assolutamente lecita. *(Applausi siamo d'accordo affinché le votazioni proseguano domani mattina, vista l'ora e la convocazione della Giunta per il Regolamento, che non ha all'ordine del giorno tale questione, ma altri rilevanti temi che da tempo il nostro Gruppo

e lo farà domani mattina.